fortemente condivisi e molto attesi dai Comuni italiani, che, come sappiamo, nella maggior parte sono di piccole dimensioni. Infatti, nei 5.585 piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti, che comprendono circa il 57 per cento del territorio italiano, vivono attualmente oltre 10 milioni di italiani. In questo contesto vi sono insediate circa 400.000 imprese agricole, impegnate ad assicurare la salvaguardia delle colture tradizionali, il mantenimento delle tipicità alimentari, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e dagli incendi. I Comuni sotto i 5.000 abitanti coprono un territorio dove, grazie all'agricoltura, si coltiva oltre la metà della produzione agroalimentare nazionale, che ha reso celebre il *made in Italy* nel mondo. Un patrimonio che fonda il suo successo anche sul terreno particolarmente fertile che offrono i piccoli Comuni alle produzioni di qualità: nel territorio di 3 piccoli Comuni su 4 sono presenti allevamenti destinati a produrre formaggi o salumi italiani DOP, mentre nel 60 per cento dei piccoli Comuni si trovano gli uliveti dai quali si ottengono i 38 oli italiani a denominazione di origine. Comuni e territori dove quest'anno si è registrato il più 76 per cento di presenze turistiche. Anche per questi dati, i piccoli Comuni sono una risorsa e non un problema per il nostro Paese. Lo stesso presidente Mattarella non ha mancato di ribadire in più occasioni che il principale antidoto all'abbandono e allo spopolamento dei piccoli territori è il rilancio della strategia delle aree interne. E tale rilancio passa necessariamente attraverso iniziative normative come questa oggi al nostro esame, volte specificamente a fissare principi di accesso ai servizi anche nuovi per quei territori, a contrastarne l'abbandono, lo spopolamento e i disagi naturali e a prevenirne il dissesto idrogeologico. Durante l'esame di merito la Commissione, pur non apportando modifiche al testo per accelerarne l'approvazione in Aula, ha voluto approvare alcuni importanti ordini del giorno che ci tengo a richiamare per temi. la distribuzione farmaceutica facilitata e l'erogazione di ulteriori servizi da parte delle farmacie medesime. Due ordini del giorno riguardano l'inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni anche degli interventi strettamente connessi alle aree in dissesto idrogeologico, di miglioramento boschivo e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, in tal senso autorizzando i Comuni a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricolo-forestali del territorio. ha ad oggetto l'estensione nel prossimo provvedimento utile delle medesime misure di questo disegno di legge anche ai Comuni sino a 10.000 abitanti. Un altro ordine del giorno è finalizzato ad assumere ogni provvedimento utile a garantire l'armonizzazione della normativa in materia di contratti pubblici con la normativa speciale a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale e per le zone montane. Anche dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sono venute indicazioni utili affinché venga valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nel procedimento di adozione dei provvedimenti di selezione dei progetti presentati, di cui parlerò a breve. Venendo alla descrizione del testo, di cui mi occuperò per la prima metà degli articoli, l'articolo 1 enuclea le finalità della proposta di legge, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Esse consistono nel favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, nel promuovere l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali Comuni, e nell'incentivare la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il disegno di legge indica altresì la finalità di favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento al sistema dei servizi essenziali e con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. La definizione di "piccolo Comune" viene ancorata, in una prima parte, alle caratteristiche dimensionali del Comune, che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Si richiede poi, in aggiunta, che il Comune rientri in una delle tipologie indicate, affinché possa beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. Il provvedimento definisce lo strumento per stabilire, rispettivamente, i criteri per la definizione dei parametri relativi alle tipologie di piccoli Comuni e l'elenco dei piccoli Comuni ai fini dell'applicazione delle previsioni normative introdotte. Si prevede per quest'ultimo elenco l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata, con un aggiornamento a cadenza triennale. Inoltre, si stabilisce che le Regioni possano definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla proposta di legge in esame per il raggiungimento delle finalità indicate, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando agli enti indicati la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali nei piccoli Comuni con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali, nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. al 2023. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse è prevista la predisposizione di un piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. In materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi, l'articolo 4 prevede la possibilità, per i piccoli Comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale L'articolo 5 consente ai piccoli Comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale, di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente poi ai piccoli Comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori. L'articolo 7 attribuisce ai piccoli Comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultralarga, stabilendo che le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si prevede, inoltre, che i progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*.

Mi consenta intanto di salutare il Governo, il sottosegretario Barbara Degani, che ci ha assistito in Commissione nel corso della discussione.

e travagliato, che ci auguriamo oggi vedrà la luce, dopo che per ben quattro volte, in quattro legislature, era approdato in Aula alla Camera senza esito. È un progetto di legge che - è bene precisarlo - non ha per oggetto il riordino istituzionale. Vi sono altri percorsi, molti dei quali incompiuti, che si occupano di questo aspetto e che vanno ripresi e completati. Essi vanno nella direzione del superamento della frammentazione e della accelerazione dei processi di cooperazione tra Comuni. Questo disegno di legge si occupa, piuttosto, di altro, come ha detto il collega Vaccari. Si occupa dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che rappresentano un segmento molto rilevante del nostro Paese.

poco meno del 10 per cento della popolazione totale del Paese. Milioni di abitanti che vivono in zone rurali, in zone interne, in aree montane, spesso ignorati da un Paese disattento, che dimentica le caratteristiche, le fondamenta, la base sulla quale l'Italia è costruita. Territori che forse rappresentano una Italia minore: piccole comunità locali che custodiscono l'identità del nostro Paese. Comunità locali con grandi storie e tradizioni che, però, ormai si sentono abbandonate e prive di futuro a causa dell'elevata età media degli abitanti e di uno uno spopolamento ingravescente. Anche se ci incoraggia il dato per cui, in questo universo di piccoli Comuni, ve ne sono tanti che negli anni più recenti sono tornati a crescere e che dimostrano che, se si attuano adeguate politiche di sviluppo locale e territoriale, questi Comuni possono avere un futuro roseo. Ecco, quindi, quanto diventa importante per questo Paese affrontare una sfida difficile, ma necessaria. Ridurre i divari territoriali, non solo tra Nord e Sud, ma anche tra Città metropolitane e periferie, tra i centri urbani e le zone rurali. Proseguendo l'illustrazione del provvedimento, riprendo dall'articolo 9 del disegno di legge, che è volto a favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi e di tariffe per i servizi pubblici erogati (acqua, gas, energia elettrica). stabilisce che nei piccoli Comuni è consentito il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari delle agenzie delle dogane e dei monopoli per l'attività di incasso e trasferimento di somme. Inoltre, si consente ai piccoli Comuni, di intesa con la Regione interessata e sulla base del contratto di programma tra il MISE e il fornitore del servizio postale universale, di proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali. Tali ambiti saranno individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali da perseguire anche attraverso il ripristino di uffici dismessi. Infine, si riconosce ai piccoli Comuni la facoltà di stipulare apposite convenzioni di intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste Italiane SpA, affinché i pagamenti relativi alle imposte comunali e ai vaglia postali possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale. Tali Comuni potranno anche affidare a Poste Italiane SpA la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. L'articolo 10 prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di una intesa tra Governo, Associazione nazionale dei Comuni italiani (l'ANCI), la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana onde adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli Comuni. L'articolo 11 stabilisce che i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Questi ultimi sono quelli il cui luogo di produzione, coltivazione o allevamento della materia prima sia situato entro 70 chilometri da quello di vendita e per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto. Nei bandi di gara indetti dai piccoli Comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di tali prodotti, inclusi quelli biologici e, in tal caso, l'utilizzo dei prodotti deve essere adeguatamente documentato. L'articolo 12 prevede che i piccoli Comuni destinino specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, sulla scorta dell'esperienza del mercato del contadino, riservando prioritariamente i posteggi ai prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile. Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una percentuale degli acquisti a questi prodotti. Viene fatta salva, infine, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta. L'articolo 13 pone in capo ai piccoli Comuni, che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali, mediante unioni di comuni o unioni di comuni montani, l'obbligo di svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e quelle che riguardano l'impiego delle relative risorse finanziarie. L'articolo 14 prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, le Regioni e le Film Commissions regionali, predisponga iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica e culturale, che si aggancia al provvedimento che abbiamo approvato L'articolo 15 prevede che il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispone il piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative. Inoltre, si prevede che, nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica

L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, con la sola eccezione delle maggiori risorse destinate alla dotazione Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, che ammonta a circa 100 milioni di euro. L'articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni legate al provvedimento trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi Statuti. Signor Presidente, è chiaro che lo spirito di fondo di questo provvedimento è delineare nuove politiche di difesa di un patrimonio che caratterizza l'identità del nostro Paese; politiche che devono tradursi in tanti progetti concreti di recupero, valorizzazione, tutela e difesa dei piccoli Comuni, nella consapevolezza che solo attraverso queste prospettive si può sperare di invertire il lento declino di cui soffrono queste comunità, senza le quali la nostra Italia sarebbe più povera e senza identità; politiche che devono tradursi in tanti progetti concreti di recupero, di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici, di difesa del territorio, di riorganizzazione e unificazione dei servizi essenziali, di valorizzazione del patrimonio artistico. Con questo disegno di legge, quindi, noi legislatori ci aspettiamo un colpo d'ala che deve venire anche dal basso, dai territori, dalle municipalità, che adesso avranno strumenti idonei a programmare, a mettere in campo progetti di sviluppo che possano costruire nuove prospettive di benessere Con questo provvedimento, quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi (e concludo), non si vuole solo difendere una storia tutta italiana a rischio di estinzione, un piccolo mondo antico, ma si affrontano anche temi attuali e moderni, che vanno dalla difesa del suolo suolo alla *green economy*, dal rapporto tra città e aree interne al completamento della banda larga, che deve essere uniformata sul territorio nazionale. Si tratta, quindi, di un giacimento di risorse che dobbiamo valorizzare e che può diventare un'occasione di crescita per il nostro Paese. È un passo forse non decisivo, ma sicuramente importante per avviare una strategia di rilancio di ciò che il presidente Ciampi chiamava la piccola, grande Italia.

Signor Presidente, i piccoli Comuni italiani, ossia le realtà amministrative con popolazione inferire a 5.000 abitanti, rappresentano circa il 70 per cento dei Comuni italiani e governano oltre il 55 per cento del territorio nazionale. Solo da questi due dati possiamo subito capire l'importanza e il valore di queste piccole realtà amministrative. L'Italia è fatta da piccoli Comuni poco visibili, ma ricchi di saperi e innovazione, caratterizzati da una forte coesione e identità sociale che si fa custode di antiche tradizioni e che costituiscono una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni. È il lavoro degli uomini e delle donne di queste piccole comunità che ha permesso di ottenere un paesaggio agricolo e ambientale di inestimabile valore e bellezza come quello italiano. piccole comunità, che spesso racchiudono il meglio della qualità manifatturiera, agroalimentare, storico-artistica e intellettuale, negli ultimi anni hanno resistito alla crisi economico-sociale che ha colpito l'Italia e l'Europa. La crisi più dura dal dopoguerra ha provocato lo spopolamento dei piccoli centri a vantaggio dei grandi poli urbani e, conseguentemente, l'abbandono progressivo di alcune parti del nostro Paese. Per questo è necessario oggi prevedere strumenti legislativi a supporto di queste comunità e, in questo senso, va la norma che stiamo per approvare. La norma mira a promuovere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, a garantire l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in essi. Non Non ci dimentichiamo che spesso chi risiede nei piccoli centri lo fa per scelta e, considerando i benefici positivi che si generano per la collettività, è giusto prevedere strumenti normativi a sostegno. I piccoli Comuni governano il 55 per cento del territorio e, oltre a rappresentare un serbatoio di biodiversità e manutenzione del territorio, rappresentano uno straordinario laboratorio di inclusione sociale e nuova cittadinanza. Molto spesso questi centri si contraddistinguono per un *welfare* di prossimità fatto di mutualità tra cittadini che collaborano tra di loro per superare i disagi quotidiani; comunità tutt'altro che chiuse dove l'inclusione e la collaborazione sono valori imprescindibili. In questa direzione vuole andare la misura legislativa che stiamo discutendo, nella quale i piccoli Comuni sono considerati risorsa per l'Italia del futuro e con la quale si prevedono misure atte a garantire, a queste comunità, servizi indispensabili come sanità, trasporti, istruzione e servizi postali. Per dare una reale possibilità di sviluppo a questi centri è ormai strategico pensare a progetti capaci di mettere in «comunicazione» piccoli e grandi centri attraverso infrastrutture moderne e integrate con il territorio. reti capaci di mettere in collegamento città e piccoli borghi, centri storici e periferie; solo così saremo in grado di garantire un modello di sviluppo al passo con la modernità, dove il telelavoro è una possibilità reale in questi Comuni. Per questo accolgo con soddisfazione i finanziamenti previsti da questa norma che mirano a migliorare le infrastrutture stradali e a portare la banda larga anche in questi territori. Ci tengo a sottolineare che questa norma prevede, tra l'altro, che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possano definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità indicate. In questo senso mi auguro che, così come molte Regioni stanno già facendo, anche le altre si attivino per prime in questa

un provvedimento che mette al centro dello sviluppo le piccole comunità, permettendo loro di continuare a svolgere al meglio il lavoro di custodi del patrimonio culturale e ambientale italiano.

dal recupero dei centri storici, andando ad acquisire gli immobili vecchi e abbandonati. E tutti sappiamo quanto, soprattutto nei Comuni più piccoli, l'abbandono o il passaggio di generazione e la stessa emigrazione dei propri dei propri abitanti abbiano portato uno spopolamento che corrisponde, nella maggior parte dei casi, anche a una fatiscenza dei centri storici. Dove non ci sono le risorse

si trovano invece delle opportunità per riattivare anche i sistemi di comunicazione e garantire ai concittadini che vivono nei piccoli Comuni i mezzi d'informazione. Penso anche

Ho presente queste circostanze nelle valli lombarde, salendo verso la montagna. Penso alla mia provincia di Varese, quando si sale in Valcuvia. Penso a Rancio Valcuvia, a Cunardo e altri piccoli Comuni che si trovano nell'alto varesotto:

Presidente, le è nota l'esperienza, che anche lei ha fatto nei giorni scorsi, recandosi a Castelluccio di Norcia. Abbiamo percorso decine e decine di chilometri senza rete Internet e senza nemmeno la comunicazione telefonica, intere vallate totalmente precluse dalla comunicazione. Chiedere alle popolazioni di quelle terre di rimanervi ad abitare, soprattutto alle nuove generazioni, è un'impresa assai ardua rispetto alle comodità e alle facili opportunità offerte dai grandi centri urbani.

circa 5.583 Comuni, che corrispondono, più o meno (per i dieci milioni di abitanti coinvolti), ad 1,40 euro all'anno per abitante per ciascuno dei Comuni o, se vogliamo sommarli nei sette anni, a circa 10 euro ad abitante. un'inezia. Se a un Comune vengono dati gli strumenti per poter procedere anche a piani di acquisizione degli immobili, si parla di svariate decine di milioni di euro per ciascun Comune.

moltissime risorse, per decine di miliardi, perché bisognava ricostruire tutte le nostre città, e soprattutto i borghi più piccoli, che sono quelli più soggetti a spopolamento e a degrado, i quali, qualora dovessero essere colpiti da un terremoto - come abbiamo visto negli ultimi giorni - difficilmente verrebbero riabitati e ripopolati, se non ricostruiti ad arte.

C'è però ancora un'altra stravaganza che mi preme mettere in evidenza, signor Presidente. Ci sono dei disegni di legge presentati da senatori e deputati del Partito Democratico

Personalmente, come la mia parte politica, sono sempre stato a difesa delle identità locali, che sono quelle che ci caratterizzano,

avrebbe dovuto essere la riforma delle Città metropolitane, che non è poi andata realmente a buon fine. Aggregare un Comune di 100.000 abitanti a una grande Città di un milione di abitanti può avere un significato molto maggiore, in termini di risparmio di risorse,

sarà, ci ritroveremo con queste poche risorse addirittura assorbite da qualche Comune privilegiato, perché nella buona manica di qualcuno che sta al Governo, lasciando a secco tutti gli altri Comuni, che non vedranno neanche il famoso 1,40 euro per abitante.

fanno un intervento non solo di estrema intelligenza amministrativa, ma anche di grande razionalità, perché riescono a offrire di più, garantendo i loro cittadini. È infatti evidente che Comuni con 200 o 500 abitanti non possono aspettarsi di riuscire a garantire servizi sociali come quelli che spesso sono necessari proprio in quei Comuni dove la vetustà abitativa normalmente è assai più alta della media italiana, perché - lo sappiamo - lo spopolamento li ha riguardati proprio direttamente. disagio insediativo, l'indice di vecchiaia, la presenza di parchi, le lacune sui servizi sociali e l'inadeguatezza complessiva dei servizi sono il *focus* del disegno di legge in esame. E tante sono le opportunità, che non voglio leggere, perché sono già state assai ben definite dai due relatori che mi hanno

provvedimento trova Comuni capaci di fare squadra - e qui, come avviene per i progetti europei, che sono quelli che stanno dando le rese maggiori, maggiori, c'è la possibilità di mettere insieme pubblico e privato, che è altra grande cosa, persino per recuperare edifici di culto o ecclesiali dismessi

L'altra questione è relativa ai tempi rapidi: abbiamo centottanta giorni, nonostante tutti i Ministeri coinvolti, per creare il Piano nazionale di riqualificazione dei piccoli Comuni. Vi

Signor Presidente, riprendo da dove ha concluso la collega. Effettivamente serve molta fantasia perché, per usare una norma che possiamo definire solo di principio che lascia poi tutti relativamente a piedi, ci vuole molta, molta fantasia.

dichiarazioni d'intenti, con la totale incapacità di risolvere minimamente il problema. Come avete già detto, si tratta di un provvedimento che potrebbe interessare il 70 per cento dei Comuni italiani, cento dei Comuni italiani, che sono sotto la soglia dei 5.000 abitanti. Chi vi parla vive in una realtà ancora più polverizzata, dove l'88 per cento dei Comuni è sotto i 5.000 abitanti. Per il Trentino-Alto Adige e per altre realtà orograficamente molto simili alla nostra, si sta parlando di sopravvivenza di un sistema sociale,

con i parametri che vengono fissati in legge, potrebbe essere penalizzato, trovandosi in situazioni forse un tantino migliori rispetto a quelle di altri Comuni. Voglio puntualizzare un'altra questione per parlare dei Comuni di montagna: quando si fissano le tipologie dei Comuni per avere titolo ad accedere ai finanziamenti,

Abbiamo posto degli *standard* basati su valutazioni squisitamente politiche. Sotto certi *standard*, il Ministero dell'istruzione ha stabilito che la scuola deve essere razionalizzata, si deve spostare un plesso da un Comune all'altro, per tutti i servizi sociali come asili, scuole materne e quant'altro. Cosa ha significato standardizzare con un parametro di livello nazionale?

Manca la popolazione, manca la domanda interna e anche le attività commerciali non ce la fanno; il negozietto che viveva a fatica finisce per chiudere.

la montagna cambia dimensione, cambia aspetto. Quei quattro anziani, a questo punto, devono essere aiutati, quasi come quando d'inverno

ai caprioli, perché altrimenti ci sarebbe una moria e conteremmo le carcasse nella primavera successiva. Bene: noi dovremo portare i servizi sociali per mantenere una popolazione

Ricordiamo che chi vive in montagna per lo più, al di là dell'attività agricola, vive anche di immagine, vive di turismo e di ambiente. Ma, se le persone non ci sono, anche la cartolina cambia, l'attrattività cambia; non c'è più attività economica e turistica.

Vengo a un altro esempio. Noi diciamo che i Comuni possono promuovere una serie di servizi essenziali, tra cui i servizi postali.

Se i quattro vecchi che vivono ancora in montagna non possono neanche andare a ritirare la pensione - l'ufficio postale alla fine serve per pagare le bollette, per ritirare la pensione e per poco altro - allora mettiamoci d'accordo.

Andiamo avanti: i piccoli Comuni possono anche istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi. Vivaddio: fermiamoci. Non facciamo fare al pubblico ciò che non sa fare.

il senatore Candiani e come avete ricordato anche voi, qua si vogliono fare le nozze con i fichi secchi: 10 milioni, che diventeranno negli anni successivi 15 milioni all'anno. È molto interessante dire che i Comuni possono acquistare immobili e riqualificarli, per contrastare l'abbandono. Una delle cose più importanti è l'abbandono del sistema turistico: l'albergo non ce la fa e chiude. Ma, se noi abbiamo 10 o al massimo 15 milioni all'anno, quante strutture alberghiere potremo comperare, acquisire e valorizzare per mantenere ancora un po' economia sui territori? Ripeto: 10 o 15 milioni all'anno. Potremmo acquistare una o due strutture. Ma stiamo parlando di una legge che va a toccare 5.600 piccoli Comuni. Non possiamo dire che risolviamo il problema

per mantenere le comunità in montagna e i piccoli Comuni, non servirebbero neanche soldi, ma servono azioni. E la Lega nel tempo ha presentato un'infinità defiscalizzare e semplificare. Una piccola attività in montagna ha più costi per la gestione del fisco che utili a fine anno. Cancelliamole i costi:

In montagna vivono per lo più agricoltori, allevatori e contadini e fanno fatica. Una cosa è fare agricoltura in pianura, grandi aree e grandi ottimizzazioni di spesa, e un'altra è farla sui gradoni, dove il prodotto è minore, la fatica è maggiore, i costi sono di gran lunga superiori e i prezzi a volte non sono remunerativi.

regimazioni delle acque sulle strade forestali»; si tratta di piccole canalette che portano via l'acqua, evitano che gli scrosci distruggano le strade e quant'altro. Un muretto di sassi, per lo più a secco, riesce a farlo anche il contadino: lo fa a casa sua e lo potrebbe fare anche per la comunità. lo sgombero della neve, tutti i contadini hanno un trattore e portano via la neve dalle aree di produzione. Allora dategli l'incarico di pulire le strade di montagna. Aiutiamoli a integrare quel reddito che oggi è insufficiente.

mano, cerchiamo di fare leggi ragionevoli che tengano in considerazione il contesto in cui saranno applicate. Se

approda qui in Senato questo importante disegno di legge. Ringrazio i relatori, il Presidente della Commissione e tutti coloro che si sono impegnati per arrivare qui in Aula e, soprattutto, i colleghi della Camera che sono entrati nel merito. un provvedimento importante, di forte carica simbolica, ma anche di norme concrete. Sarà insufficiente, senz'altro. Intanto, però, si inizia. Altri, prima di noi, avrebbero potuto farlo e non lo hanno fatto. giunge, peraltro, a un anno di distanza da un drammatico terremoto che ha colpito proprio una parte di Appennino costituita da una miriade di piccoli Comuni. legge stanzia cento milioni, che poi aumenteranno nel corso degli anni, e ha lo scopo di risollevare le sorti dei piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti. Così come è già stato detto - e lo ripeto - solo 5.585 Comuni, pari al 70 per cento del totale dei Comuni presenti sul territorio italiano; oltre 10 milioni di cittadini italiani che comunque, nonostante le difficoltà, continuano a risiedere in questi territori. È una legge molto attesa, è una opportunità per l'Italia, ha una forte innovazione ed è in controtendenza rispetto a politiche di altri Governi, punitive verso le piccole realtà. Dietro questa iniziativa c'è un pensiero forte, che viene da lontano, che ha visto generazioni di giovani, di intellettuali e di ambientalisti interrogarsi sul futuro di questi territori; che ha visto miriadi di sindaci, nel corso degli anni, impegnarsi e mobilitarsi. Io mi sono battuta per anni contro l'abbandono, la chiusura dei presidi territoriali, la mortificazione dei territori e la mortificazione di una storia millenaria, che proprio lì, nei piccoli Comuni, specie nelle nostre montagne, si concentra.

stanno qui in Senato e che allora avevano ruoli amministrativi, il progetto di Appennino Parco d'Europa, affinché montagne e piccoli centri diventassero area di sperimentazione di un nuovo sviluppo. questo oggi sono doppiamente contenta, come senatrice del Partito Democratico - un partito che le cose le dice e le fa - e come donna dell'Appennino, che può tornare a sperare, e come persona che viene da una terra, appunto, di piccoli Comuni. Emerge una idea di sviluppo che punta sui territori e sulle comunità, che coniuga storia, cultura, saperi tradizionali con l'innovazione e le nuove tecnologie, la *green economy*. una legge, questa, che aiuterà l'Italia a essere più forte e più unita. Il provvedimento nasce da una proposta di legge di Ermete Realacci che, durante l'esame a Montecitorio, è stata poi unificata ad altra legge ed è arrivata qui in Senato. L'importanza dei piccoli Comuni si è vista anche nel terremoto, con il ruolo fondamentale per la tenuta delle comunità svolto proprio dai municipi. I nostri piccoli Comuni amministrano, quindi, una parte importante del territorio nazionale. Non sono una eredità del passato, ma una straordinaria occasione per difendere la nostra identità, le nostre specialità e proiettarle nel futuro. Il disegno di legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni prevede un vero e proprio Piano Piano nazionale per la riqualificazione dei borghi con meno di 5.000 abitanti. Stanzia delle somme, che potranno certo essere aumentate, ma che non sono mai state stanziate prima, e propone anche misure per favorire la diffusione di banda larga, servizi più efficienti, itinerari di mobilità e turismo dolce. proprio al fatto che oggi a Campotosto, epicentro di recenti terremoti, parte l'itinerario del Tratturo Magno. Poi c'è la promozione di produzioni agricole e agroalimentari a filiera corta. In più, il provvedimento introduce semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono. Prevede opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell'ambiente, messa in sicurezza di strade e scuole, efficientamento energetico del patrimonio edilizio. I piccoli Comuni potranno anche acquisire case cantoniere e tratte di ferrovie dismesse da rendere disponibili per attività di protezione civile, volontariato, promozione di prodotti tipici locali e turismo. Si tratta, quindi, di una legge importante per mettere queste realtà in condizione di essere non un peso, una zavorra il nostro Paese, ma una straordinaria occasione. Molte sono le misure previste, citate anche dai relatori: si va dalla possibilità di registrare la nascita

Importante è anche la previsione del recupero dei cammini storici: sono stanziate risorse proprio per collegare i piccoli Comuni su questi antichi e storici cammini; il recupero dei borghi, con interventi antisismici, e diverse misure a sostegno dei prodotti tipici locali, come ad esempio la vendita diretta all'interno di punti commerciali, l'incentivo della filiera corta e la valorizzazione delle delle attività pastorali di montagna. Obiettivo storico è frenare il disagio demografico ed economico che colpisce oltre 2.000 piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, da cui i giovani tendono ad andare via e le case abbandonate o vuote sono addirittura una ogni tre. I piccoli Comuni detengono, tra l'altro, la gran parte del patrimonio di biodiversità agroalimentare. Vi si coltiva oltre la metà della produzione agroalimentare nazionale che ha reso celebre il *made in Italy* nel mondo, grazie alla presenza di oltre 300.000 imprese agricole. piccoli Comuni su quattro sono il territorio di riferimento per gli allevamenti destinati a produzioni importanti a denominazione di origine protetta (DOP), mentre nel 60 per cento dei borghi si trovano gli uliveti dai quali si ottengono i pregiati oli italiani a denominazione di origine protetta. Ma moltissimi, anche in Abruzzo, sono i veri e propri gioielli di produzioni tipiche e a volte i nomi i nomi dei Comuni si associano a quelli dei prodotti tipici. Vale la pena ricordare, proprio per le cose che sono state dette, che l'*iter* della legge è stato molto complicato e che altre legislature non hanno avuto la forza di concluderlo. La prima proposta di legge è del 2001 e dal 2001 al 2017 sono passati in questo Paese Governi di altra ragione politica e di altra realtà, ma che non vollero o non poterono condurre a termine questa iniziativa.

occasioni in cui fu presentato, da parlamentari di ogni parte politica ed Ermete Realacci fu il conduttore, allora, di questa battaglia, oggi diventata comune e addirittura rivendicata da chi la Comunque, ci siamo arrivati e ci siamo arrivati bene. La Camera ha approvato all'unanimità il testo e sicuramente anche in questa occasione ribadiremo quell'unanime consenso.

ma anche un impegno speciale, all'indomani dell'approvazione della legge, affinché si impostino concrete politiche attive per arginare lo spopolamento e l'abbandono del territorio. Ne avrà vantaggio tutta l'Italia, anche le aree metropolitane, che spesso

colleghi, intanto lasciatemi dire che attendere quattro legislature per tutelare le condizioni di vita di 5.585 piccoli Comuni italiani è vergognoso. Lasciatemi anche aggiungere che non è semplicemente una questione di numeri.

il loro fondamento in quella biodiversità che ha voluto offrire nel nostro territorio, anche da un punto di vista propriamente geografico, demografico e antropologico,

Attendere cinque legislature per ottenere una legge a tutela di queste realtà è qualcosa di vergognoso che ricade sulle forze politiche che hanno deciso, essendo maggioranza nei precedenti Parlamenti, di dimenticare tutto ciò. E lasciatemi aggiungere un dato. Se è vero che noi ogni anno malediciamo terremoti e la senatrice Pezzopane ricordava che l'anno scorso eravamo tutti impegnati a fronteggiare l'ennesima scossa tellurica che aveva funestato in particolar modo il Centro Italia, se è vero che ogni anno dobbiamo far fronte ad alluvioni, a tracimazioni, e esondazioni, a frane e smottamenti che hanno un costo, prima prima ancora che economico, in termini di vite umane, di danni all'ambiente e di emotività danneggiata,

i processi di inurbamento della popolazione italiana non vanno semplicemente subiti e non vanno neanche governati, ma vanno ostacolati quando sono assolutamente dissennati. allora coscienza, come ribadiscono ormai tanti antropologi, tanti demografi e geografi, che una popolazione concentrata soprattutto su realtà urbane particolarmente consistenti è un danno per l'ambiente tutto e per la popolazione stessa in termini di qualità della vita, se è vero che tutti quanti ci riempiamo la bocca di quei piccoli borghi in cui, come diceva la senatrice Pezzopane, dobbiamo andare a passare i *weekend*. Ma perché dobbiamo passarci il *weekend*? E poi, scusatemi, perché non recuperare la tradizione della nostra lingua: perché non passarci il fine settimana? O, aggiungo, perché non viverci stabilmente? Questo dipende dalla politica, perché se tu quei piccoli centri li abbandoni e quindi pregiudichi la sopravvivenza dei servizi essenziali, allora una tua responsabilità in quanto forza di Governo c'è. Pongo allora una domanda a tutti. L'Italia è un Paese che contempla al suo interno, soprattutto al Nord, una pianura rilevante che conosciamo tutti e chi presiede appartiene a una forza politica che della Padania ha fatto il suo epicentro simbolico, però l'Italia è soprattutto montagna e collina, che è stata nel tempo antropizzata con difficoltà. Prima il senatore Divina, che adesso manca, faceva riferimento, per esempio, ai terrazzamenti con cui generazioni di contadini hanno assoggettato all'agricoltura dell'uomo gole, valli e territori comunque scoscesi e impervi, ottenendo produzioni di ottimo livello e qualità e questo sia al Sud, che al Centro, che al Nord. Dopo la Seconda guerra mondiale, abbiamo seguito alcuni miti consumistici e americaneggianti invece della nostra civiltà di riferimento, che era essenzialmente una unità contadina, in cui i valori di comunità erano

che l'Italia è costituita da circa 8.000 Comuni e che, quindi, in termini di centri che conservano una loro identità, una loro storia e una loro proposta come *ratio essendi* per sopravvivere anche nel XXI, XXII e XXIII secolo, c'è tanto e se noi accettiamo, per esempio, che vi sia una svalutazione del patrimonio immobiliare di questi piccoli borghi, colpiti da una fiscalità assolutamente irrazionale ed iniqua, noi decretiamo la fine di quei centri. E allora questo era un provvedimento centrale, ancor più delle varie leggi che arrivano e in quattro e quattr'otto vengono approvate perché bisogna portare fieno in cascina ai partiti e ricordiamo tutti a cosa faccio riferimento: ad esempio, alla cosiddetta la leggina che ha permesso ai partiti di portare nel cassiere subito, *cash*, oltre una quarantina di milioni di euro. Addirittura una quarantina di milioni di euro subito, quando chi chi mi ha preceduto ricordava che questo provvedimento stanzia negli anni, non immediatamente, 100 milioni di euro. Una cifra enorme!

Noi, come ovvio, rimarcando tutte queste criticità, non possiamo tirarci indietro e quindi voteremo a favore del provvedimento perché finalmente è qualcosa. Ed è qualcosa - e qui faccio una notazione di merito e di metodo - anche perché alla Camera, dove il provvedimento si è incardinato, si è deciso da parte del partito di maggioranza relativa di dialogare

parti importanti di un'altra proposta di legge promossa in particolar modo da Patrizia Terzoni come prima firmataria e dal Movimento 5 Stelle tutto. tutto. Attraverso un dialogo che è stato difficile, ma comunque costruttivo, qualcosa è stato recepito, ma "qualcosa" è ancora ben poco rispetto a quello che quegli italiani debbono giustamente vedersi riconosciuto.

dopo la pensione, chi ha vissuto tutti i suoi anni migliori a Roma, a Firenze o in qualche altra grande realtà urbana, possa andare a recuperare la qualità della vita in Provincia di Sondrio, di Cosenza di Cosenza o di Caltanissetta, magari in un borgo che offra come valori immensi, per esempio, la qualità del pane oppure la straordinaria suggestione di un paesaggio. Certe volte, quando si osserva la natura, senza scomodare i grandi, ci si rigenera. E certamente questa capacità non la offre la grande metropoli o la megalopoli: nel caso, quella offre qualche mesotelioma, qualche problema oncologico relativo all'inquinamento in cui si è costretti a vivere. a vivere. Ribadendo le parole di Arminio, noi vorremmo che in questo Paese si promuovessero stili di vita per cui non si va a terminare la propria esistenza nel piccolo borgo, ma si accompagna tutto il proprio vivere in quelle strade, in quei luoghi, in quei posti che hanno permesso, ad esempio, a uno dei più grandi maestri della poesia italiana, Giacomo Leopardi (ieri in quest'Aula ricordavamo dei grandi della nostra cultura) di rendere universali borghi che altrimenti potevano essere conosciuti soltanto da chi vi viveva. però è un problema di atteggiamento mentale, di cultura, di mentalità. E voi che mentalità avete, se solo e soltanto promuovete la realizzazione di centri commerciali? Perché ieri è stato un sindaco di Forza Italia? Semplicemente perché aveva favorito l'ennesimo centro commerciale che indirettamente facilita lo svuotamento delle valli, delle colline e delle montagne per favorire chi sta in pianura e questa è la politica che voi, dissennatamente e in maniera anche funzionale

deve, ad esempio, puntare sulla montagna, sulla collina, su queste realtà per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per un rilancio di attività produttive realizzate con creatività, con fantasia, perché la maestria di un maestro impagliatore o di un liutaio nessun *robot*, nessuna stampante in 3D la potrà garantire. Tuttavia, per far questo non sono sufficienti 100 milioni: è l'inizio e la prossima sfida dei prossimi Parlamenti sarà quella di ostacolare le leggi Boccadutri e di favorire leggi che abbiano anche come primo firmatario un esponente non del Movimento 5 Stelle, ma che abbia a cuore le esigenze e i diritti reali degli italiani.

al coro dei colleghi del Partito Democratico che mi hanno preceduto, perché io ci vivo in un piccolo Comune dell'entroterra del Sud, pur non essendo ancora arrivata all'età della pensione e quindi tengo a sottolineare l'importanza del disegno di legge in esame, che pone un cambiamento di marcia completo rispetto a quanto in passato è stato fatto (o meglio non fatto) per queste aree. Si tratta di un piccolo passo per valorizzare le piccole realtà, per migliorare le condizioni di vita in queste aree, acquisendo finalmente la consapevolezza delle risorse e delle potenzialità che le nostre aree interne hanno, come è stato detto, da tutti i punti di vista (culturale, sociale, ambientale e delle produzioni tipiche locali). Dunque finalmente i centri minori tornano protagonisti e al centro del dibattito politico, dopo che erano rimasti per troppo tempo ai margini del dibattito pubblico.

dei servizi essenziali per i cittadini. Abbiamo già detto che su 8.000 Comuni italiani 6.000 hanno popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, quindi ci stiamo rivolgendo a una parte molto rilevante del nostro Paese. I circa 6.000 Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti non sono soltanto una priorità dal punto di vista numerico,

di riduzione dei costi, senza pensare alle difficoltà ed alle maggiori necessità che questi Comuni hanno proprio per il disagio in cui vivono. Aggiungo, peraltro, che, al contrario, l'equilibrata distribuzione della popolazione sul territorio va a garanzia di tutto il sistema sociale e culturale del Paese, non soltanto a beneficio e a vantaggio di queste piccole realtà e faccio riferimento, in particolare, alle questioni già sollevate della manutenzione del territorio e del patrimonio, del patrimonio, del grande apporto che questi Comuni possono portare all'equilibrio del Paese. L'obiettivo che questo disegno di legge si pone, quindi, è sicuramente apprezzabile. arriva con un po' di ritardo, ma finalmente arriva, e arriva in questa legislatura e si aggiunge agli altri provvedimenti che in questo periodo sono stati messi in campo a favore di queste piccole realtà e della costruzione di un sistema che miri a creare le condizioni perché i nostri giovani possano continuare a vivere dignitosamente nei piccoli paesi e nei luoghi dove sono nati.

Cominciamo così ad agevolare le iniziative economiche e commerciali dei piccoli imprenditori che vivono in quei Comuni e che molto spesso sono veramente sopraffatti e soffocati. Anche l'iniziativa privata del ragazzo che vive nell'area interna di un piccolo Comune spesso è soffocata dagli interminabili *iter* burocratici e dal doversi districare in condizioni davvero complicate. È importante evidenziare, tra le priorità che il fondo prevede, anche il recupero e la riqualificazione urbana dei centri storici, dei terreni, degli edifici in stato di abbandono.

Italia. La maggior forza per i piccoli Comuni non deriverà quindi da operazioni artificiose, ma potrà discendere da una rinnovata consapevolezza delle proprie possibilità e della propria dignità, che vuol dire anche valorizzazione della propria storia e delle proprie tradizioni. La rinascita dei territori non può venire dall'acquiescenza alle politiche di bilancio che privilegiano i grandi centri, ma soltanto da un nuovo investimento in termini di energie, da mettere il più possibile al servizio di processi virtuosi di crescita programmatica e partecipata. Infine, un'ultima piccola annotazione: i piccoli Comuni sono numerosi, se rapportati al complesso degli enti locali esistenti nel nostro Paese, e e costituiscono l'articolazione tipica del nostro Centro Sud, un'area che è stata fortemente colpita dalla crisi degli ultimi anni, che ha necessità di particolare attenzione per poter

È un provvedimento che affonda le radici - com'è stato detto nei tanti interventi dei colleghi che mi hanno preceduta - nella storia del Paese

può facilmente dirsi anacronistica per l'insostenibilità da parte di molte municipalità italiane dell'erogazione di servizi, a causa della ridotta dimensione, spesso solo demografica e non territoriale, del Comune,

sempre maggiori, sia in essere, sia in divenire. Per far fronte a questi problemi la strada della razionalizzazione degli enti locali, ha spinto, spinge e sta spingendo verso fusioni e unioni territoriali intercomunali.

la mia Regione, sta sperimentando, non senza problemi e necessità di correttivi, le unioni territoriali intercomunali (UTI). I contenuti del provvedimento, tuttavia, non affrontano il tema della riorganizzazione dell'ente locale, bensì intervengono nella difesa e nella valorizzazione dei territori e delle comunità dei piccoli Comuni, che vogliono e devono mantenere le proprie peculiarità e non rinunciarvi, né in parte, né *in toto,* e non solo in una logica di sopravvivenza, ma in una logica di rilancio. Si guarda alla tutela di quei territori e di quelle comunità che rischiano di chiudere a causa dell'abbandono delle abitazioni per trasferimenti lavorativi (ne sanno qualcosa

di piccoli ma importanti aiuti, grazie ai grandi finanziamenti che qui sono previsti, attraverso i quali rilanciare il ripopolamento di queste aree e di queste comunità che che vogliono rimanere tali e non intendono rassegnarsi a divenire territori abbandonati e comunità atomizzate in via di estinzione. Si richiedono, perciò, sostegno e riqualificazione per questi Comuni: difesa del suolo, *green economy*, misure di contrasto all'abbandono e supporto alle esigenze anche dell'edilizia scolastica.

3 compare un elenco di interventi prioritari che devono mirare alla riqualificazione e manutenzione del territorio, alla messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici

(la filosofia della *green economy*, appunto), dell'acquisizione e riqualificazione di terreni ed edifici in stato di abbandono, sedimi ferroviari e via dicendo. Lungi dal ritenere questo aiuto un mero strumento di assistenzialismo statale, le comunità dei piccoli Comuni oggetto del provvedimento dovranno fare la loro parte.

Questo è l'apprezzabile spirito del provvedimento in esame, che vuole rivolgere attenzione alle esigenze insopprimibili delle numerose piccole e preziose comunità del nostro Paese.

XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento in esame proviene dalla passata legislatura quando, strombazzato ai quattro venti dal duo Lupi-Realacci, è finito nel cassetto stante la sua inutilità. Si tratta di una minestra riscaldata che ci viene servita in questa legislatura, insignificante, inadeguata e inutile. Un provvedimento che non serve a niente, fumo negli occhi per ignari cittadini che non conoscono la realtà delle cose. Sappiamo bene che idea avete delle autonomie locali. Alle autonomie locali voi preferite il centralismo democratico. Ma voi conoscete i problemi dei Comuni italiani, degli oltre 5.600 Comuni con meno di 5.000 abitanti? Onestamente non sono affatto sorpreso. I vostri pensieri sono mal celati. Conosciamo bene quali sono i vostri obiettivi: distruggere gli enti locali. Prima avete massacrato le Province, ridotte a enti di secondo grado, grado, privato i cittadini della possibilità di scegliere i loro rappresentanti di area vasta, ridotto le competenze e il personale effettuato tagli feroci delle risorse, tanto che le Province non sono in grado di poter adempiere neanche minimamente alle quattro funzioni che sono ancora rimaste di loro competenza: scuola, viabilità, ambiente e urbanistica. stato fatto in aperta violazione della Costituzione. Tanto per voi la Costituzione, le leggi e i regolamenti sono carta straccia, *optional*. Adesso la vostra azione prosegue portando i Comuni al dissesto e al fallimento, tagli alle risorse e al personale e adempimenti burocratici continui e asfissianti, condannandoli così a una lenta e inesorabile agonia. Il vostro disegno è chiaro. D'altra parte, è scritto

modifica al testo unico del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di popolazione dei Comuni e di fusione dei Comuni minori. bisogna trovare un efficace meccanismo per ridurre la frammentazione dei Comuni italiani: bisogna cioè distruggere comunità con 1.000 anni di storia; ovviamente, tutto questo con la complicità dell'ANCI, altra associazione del tutto inutile, che brucia denaro pubblico in quantità industriale. Gli oltre 5.600 Comuni sotto i 5.000 abitanti devono sparire con il pretesto del miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Ma perché non pensate a migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi nei Comuni più grandi, dove il loro costo per abitante per abitante è spropositato e lo sperpero di denaro pubblico, le ruberie e il degrado riempiono le pagine dei giornali tutti i giorni? C'è di più, voi siete capaci di fare altro. Vi racconto cosa sono stati capaci di fare nelle Marche. Le amministrazioni e i sindaci di Serrungarina, Montemaggiore al Metauro e Saltara decisero di fare un *referendum* sulla fusione dei tre Comuni. fu la partecipazione, ovviamente: su 9.693 aventi diritto al voto, si presentarono in 2.652 a dire sì.

Accorpamento forzato: o con le buone o con le cattive, dovete fare quello che diciamo noi. Nessuno era mai arrivato a tanto, neanche nel periodo fascista: il Fascismo, quando

in cui fossero mancati i mezzi per provvedere in maniera conveniente ai servizi pubblici. Poi, nel dopoguerra, il nuovo Governo consentì la ricostruzione dei Comuni fino a 2.000 abitanti che erano stati soppressi.

Con questo provvedimento stanziate 100 milioni in sette anni: 10 il primo anno e 15 nei sei anni successivi; se ripartite questa somma su 5.600 Comuni, siamo alla ridicola cifra di 2.500 euro per ogni Comune: è una vergogna. Sono eroi gli amministratori dei piccoli Comuni che al giorno d'oggi si fanno carico di amministrare le loro comunità, schiacciati dalle responsabilità, dalla burocrazia, dai problemi e dalla mancanza di risorse. Spesso i sindaci non sanno dove sbattere la testa. I sindaci dei piccoli Comuni quando hanno un contratto di servizio a trenta giorni pagano la fattura all'imprenditore che lo svolge; non fanno come il Governo che paga dopo due anni (la pubblica o come fa il Comune di Roma, che ogni tanto fa un accomodamento e si rende necessario affidare ad un commissario la gestione separata dei debiti accumulati. sui Ministeri bisogna intervenire per tagliare la spesa e gli sprechi. Mi dovete spiegare come mai il debito pubblico, in questi cinque anni, è cresciuto di 360 miliardi mentre gli enti locali lo hanno ridotto di 7 Gli enti locali negli ultimi cinque anni hanno contribuito al risanamento dei conti pubblici per oltre 15 miliardi, magari lo avesse fatto lo Stato. Ai Comuni minori serve autonomia organizzativa, gestionale, decisionale, fiscale, impositiva. Ai Comuni serve poter fare programmazione, poter contare su risorse certe. Quando li fate voi i trasferimenti? A fine anno? Ai Comuni serve poter fare investimenti anche sulla manutenzione straordinaria. Una volta i Comuni potevano fare mutui fino ad una quota pari al 25 per cento dei primi tre titoli di entrata addirittura del bilancio preventivo, che si poteva anche un po' forzare; oggi siamo al 10 per cento dei primi tre titoli del bilancio consuntivo di due anni prima. Oggi le risorse il Governo le assegna con la demenziale modalità del *click day*, ignorando che le condizioni della rete telematica sono diverse in ogni realtà italiana e il peso dei *file*, ovvero gli allegati del progetto, incidono sulla velocità di trasferimento delle domande.

ha, in questo caso, bloccarne la sostituzione? Bisogna consentire ai Comuni di utilizzare anche quella sola figura

Bisogna semplificare la contabilità, che non può essere la stessa per un Comune di 2.000 abitanti e per un Comune di 2 milioni di abitanti. Bisogna semplificare le procedure di appalto.

a dopodomani per esprimere un giudizio assolutamente negativo su questo provvedimento, che risulta essere del tutto insignificante, inadeguato ed inutile. La montagna ha partorito il topolino, questo è il titolo che si potrebbe dare a questo disegno Per disciplina di partito, ovviamente, seguirò le indicazioni del Gruppo ma il mio pensiero è chiaro.

inserisce in un processo di razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi attraverso riforme istituzionali e cerca, allo stesso tempo, di dare valore e trovare soluzioni specifiche dedicate a quella grande parte d'Italia che racchiude in sé patrimoni unici. cerca di sostenere la "tenuta" di quei luoghi dove si producono le maggiori eccellenze agricole certificate del nostro Paese, dove il prodotto coincide con il territorio e spesso il nome delle produzioni si identifica con il nome della montagna. a quei territori di montagna in cui, nel secolo scorso, nel periodo della corsa all'industrializzazione, si è aperta una fase di spopolamento - non ancora finita - nelle zone più alte della montagna, una fase in cui si erano centralizzati nelle grandi aree urbane i servizi e le funzioni economiche e culturali, facendo diventare periferia i piccoli centri, facendo diventare marginale la cultura rurale, lontana fino al punto di perdere il rapporto tra il cibo e la sua origine, fino a creare una frattura, una dispersione di saperi e di consapevolezze sul valore della produzione alimentare. Il grande centro urbano come catalizzatore di tutto.

la produzione intensiva. Non sono d'accordo con i colleghi che mi hanno preceduto. Stiamo invertendo la rotta di quell'idea di Italia. Lo abbiamo fatto in questi anni, in questa legislatura, in particolare con le leggi che valorizzano la biodiversità: il collegato ambientale, il collegato agricolo, la strategia importante delle aree interne, con risorse mirate al recupero dei borghi. L'agricoltura, anzi le agricolture sono al centro di una nuova idea di sviluppo, di nuove professioni professioni in agricoltura per le nuove generazioni. Questo è un dato, sono fatti. Spero poi che quest'Assemblea colga l'occasione di approvare la legge sul biologico e sulla dieta mediterranea in quest'ultimo squarcio di legislatura. noi continuiamo questa sfida anche in questo provvedimento sui piccoli Comuni, per valorizzare la ricchezza delle differenze e delle varietà, il nostro primo fattore competitivo in un mondo standardizzato. Stiamo invertendo la rotta nel rapporto tra funzione dell'urbano e nuove funzioni delle aree rurali e possiamo farlo ora, in questo tempo in cui gli elementi essenziali dei cambiamenti epocali, che sono la comunicazione e la produzione di energia, non sono più fondati su sistemi centralizzati. La comunicazione è fondata ora sulla diffusione in rete e l'energia sulla possibilità di produzione diffusa. Questo cambia tutto e apre una nuova idea del vivere. Ogni punto della rete ha la possibilità di diventare un centro, se si hanno le capacità, se vi è creatività, se vi è motivazione. Servono infrastrutture e servono rapidamente. Non è un dettaglio l'articolo della legge che sostiene lo sviluppo della banda larga nei piccoli Comuni, perché questo è un elemento determinante. È una conquista di pari opportunità di comunicazione veloce, nel piccolo Comune di montagna come nella grande area urbana. È la differenza tra essere terminale e subalterno a funzioni direzionali nate altrove o essere protagonista in azioni imprenditoriali e culturali. un provvedimento che guarda dunque a quell'Italia preziosa e ricca di opportunità, ma anche altrettanto fragile, ancora a rischio di abbandono, dove la possibilità di vita della comunità e delle famiglie è legata spesso alla tenuta di una scuola, alla qualità e alla sicurezza di un servizio ospedaliero o di un punto nascita in cui il valore sanitario e il valore sociale si intrecciano. In quelle aree la permanenza dei giovani diventa precondizione per ogni altro Sì, sono importanti le risorse che vengono assegnate in questo provvedimento. Non sono abbastanza e dovranno essere certamente incrementate, ma non sono l'unico elemento importante e l'unico discrimine. Non sono d'accordo con il collega Candiani: lo stimolo è quello di rilanciare antichi patrimoni come elementi fondamentali per un'idea di futuro possibile. È una svolta culturale, è un ulteriore strumento per individuare, come viene richiamato nella legge, soluzioni inedite di servizi multifunzionali, per le poste, per la formazione, per il turismo con ospitalità diffusa. Ciò che è molto importante nella legge è che si aprono nuove possibilità che si sganciano dalla rigidità degli standard numerici come unico criterio di valutazione. Ciò che diventa davvero determinante ora è che tutto questo sia immediatamente riconosciuto, attivato e coerente con le scelte in atto, con i provvedimenti legislativi in corso. che siano riconosciute queste priorità dalle Regioni e che sia riconosciuto il senso di questo provvedimento, mentre si prendono decisioni parallele sulla tenuta dei presidi ospedalieri, sui presidi scolastici, sull'idea di sostegno all'iniziativa imprenditoriale, tenendo in conto le specificità. alle imprese agricole capaci di produrre eccellenze uniche, come imprese ad alto livello di complessità. È necessario sostenere chi affronta la sfida della produzione agricola ecosostenibile e non invece fornire un'assistenza generica e indistinta. Questo è il cambiamento. Ritengo, signora Presidente, che questo sia un salto culturale di grande importanza, un investimento sul futuro basato sul binomio di tradizione e innovazione, su soluzioni inedite da ricercare, con alcuni criteri da reinventare paradigmi da reimpostare. Siamo in una fase di transizione e, se punteremo convintamente su originalità, valore qualitativo alto, salvaguardia del patrimonio storico-culturale e ambientale,

c'è da mettersi le mani nei capelli. Se io fossi un sindaco di un Comune sotto i 5.000 abitanti o se fossi un sindaco che dovesse beneficiare di questa svolta epocale, sarei un po' arrabbiato, per il semplice motivo che questa svolta epocale,

Mamma mia, che svolta epocale! Wow, se fossi un sindaco, a questo punto stapperei lo *champagne* e direi: «Ho risolto i problemi del mio bilancio!». Andiamo a vedere questa svolta epocale in cosa consiste. All'articolo 2, («Attività e servizi») si parla di costituzione di centri polifunzionali: benissimo, una bella svolta epocale, ma con quali soldi? Con 2.500 euro all'anno facciamo dei centri polifunzionali? All'articolo 3 («Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale») mettete a disposizione ben 25 milioni di euro per 5.000 Comuni; Comuni; sembrano tanti, ma per fare che cosa? Tutela dell'ambiente, tutela dei beni culturali, mitigazione del rischio idrogeologico, salvaguardia dei centri storici, messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e scolastiche, promozione dello sviluppo economico: il tutto con 25 milioni di euro da dividere tra più di 5.000 Comuni. È una svolta epocale! All'articolo 4 («Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi») manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti, riuso del patrimonio edilizio, miglioramento degli arredi urbani, consolidamento antisismico degli edifici storici. È vero che è una svolta epocale, ma con 100 milioni di euro e 17.000 euro in sette anni per Comune, la svolta epocale è solo nella mente dei senatori del Partito Democratico.

anche questo verrà finanziato con quei famosi 25 milioni di euro di cui parlavo prima. Oltre a tutto quello che vi ho detto, c'è anche questo. Ma stiamo prendendo in giro? Se dobbiamo prendere in giro 5.000 sindaci, diciamolo.

signor Franceschini, rispetto alle case cantoniere. Si affidi a chi di turismo ne capisce. Anche in questo caso, però, non sviluppiamo il turismo con le case cantoniere a spese del Ministero del turismo, bensì delegandolo ai piccoli Comuni e dicendo ai piccoli Comuni: «Il turismo viene sviluppato con le case cantoniere

o, anche in questo caso, è il libro dei sogni, scritto così perché bisognava scrivere qualcosa, magari per tenere buoni i sindaci dei piccoli Comuni in vista delle prossime elezioni? Perché a me sembra questo. diffusione della stampa di cui all'articolo 10, siamo d'accordo, è una bellissima idea: una edicola in ogni piccolo Comune. Ma per permettere a uno di fare l'imprenditore, andare in un piccolo Comune, diffondere la stampa locale, fare l'edicolante in un momento storico in cui le edicole stanno chiudendo nei grossi centri,

Signori, ci vogliono i soldi. Caro Governo, ci vogliono i soldi per venire in Aula a raccontarci il libro dei sogni. Personalmente, a Gian Marco Centinaio sembra di essere tornato a ieri. Provvedimenti che non servono a nessuno.

È un segnale utile alle realtà delle nostre piccole comunità e, sul piano normativo, corrisponde all'esigenza di estendere poteri e opportunità per le nostre piccole amministrazioni comunali. comunali. Rimane un tema che credo che anche il relatore e lo stesso Governo si pongano: ho idea che le dotazioni finanziarie che abbiamo visto inserite nel progetto di legge

già dalla prossima legge di bilancio, intervenire su questi argomenti rafforzando sul piano finanziario le cose buone che ci sono sotto il profilo normativo. Detto questo, vorrei

vengo da una Regione che ha un indice negativo di crescita e una proiezione demografica di desertificazione antropica molto rilevante.

in meno, in una Regione che ha la bellezza di 377 Comuni (perché il territorio è vasto),

pur essendo una bellissima Regione, paga il prezzo, rispetto alla

l'insularità, interpretata in ragione dell'insufficienza dei collegamenti con le reti nazionali ed europee; un'insularità che è interpretata nel senso dell'isolamento, cosa oggi superabile, anche tecnicamente.

Non voglio qui aprire un capitolo che conosco ma non così approfonditamente come altre forze politiche di questo Senato. Mi riferisco, per esempio, allo spopolamento nelle realtà montane. Non voglio aprire questioni che si devono pure affrontare per le isole minori. Eppure anche questo è uno degli argomenti di cui dobbiamo occuparci. Neppure voglio aprire la questione che riguarda la gestione della vita delle persone, delle nostre comunità, dei gravi problemi che riguardano il lavoro e della possibilità di inserimento attivo nella società società dei nostri giovani. Questi sono però i temi da affrontare per contrastare lo spopolamento, per mantenere vive le nostre piccole comunità, perché vanno mantenute tali in ragione degli stessi obiettivi che questa legge si pone, che sono principalmente il governo del territorio, la sua manutenzione la sua difesa dai pericoli. In cosa consiste il mantenimento delle identità e delle appartenenze come radici necessarie per lo sviluppo anche delle personalità? personalità? Nella difesa del nostro immenso patrimonio culturale, archeologico e storico,

perché sta facendo una scelta di fondo insostenibile e da combattere. Esattamente si pone il problema della gestione del declino di questo Paese e ciò va evitato.

Non è accettabile che si rinunci alle opportunità che ci vengono dal mondo, dai suoi fenomeni e dalle ragioni per le quali si sviluppano processi per rafforzarci anche sotto il profilo demografico. La demografia è un dato da tenere sempre presente perché incide su tutto. tutto. Lo dico a coloro che vogliono difendere le piccole comunità salvando le edicole: per salvare le edicole bisogna che ci sia qualcuno che compri il giornale, altrimenti le edicole chiudono perché non c'è nessuno che va a comprare il giornale. Per salvare gli immobili nelle nostre piccole comunità, bisogna che ci sia qualcuno che li abita, altrimenti deperiscono, si degradano e crollano perché nessuno mantiene una casa in cui non vive: l'abbandona anche se ne è proprietario.

di occuparsi anche di settori nei quali i nostri connazionali ritengono di non doversi più impegnare. Abbiamo sei milioni di stranieri che hanno in buona parte o in parte consistente il diritto alla cittadinanza. Abbiamo giovani che qui hanno studiato e sono cresciuti; sono italiani fino all'ultima cellula della loro capacità di essere cittadini, perché questa è la condizione che hanno vissuto nelle scuole, nelle università partecipando a progetti di professionalizzazione. Abbiamo sei milioni di stranieri, molti dei quali hanno maturato, rispetto ad una logica anche giuridica

- è inter-etnico e interculturale; bisogna pertanto pensare al rispetto nei confronti di tutti e all'acquisizione del rispetto di tutti attraverso processi di integrazione vera che facciano di questa risorsa umana importantissima una leva dello sviluppo complessivo del nostro continente e del nostro Paese. Attenzione perché se non facciamo così, saremo quelli che costruendo muri, finiranno per starvi sotto, perché essi crolleranno sotto il peso di una responsabilità dovuta ad una miopia politica insostenibile. Possiamo rilanciare le nostre piccole comunità attraverso un'attenzione allo sviluppo demografico del nostro Paese. Ciò vuol dire aiutare anche le famiglie, famiglie, le giovani coppie, coloro che vorrebbero rimanere in Italia, che si sono professionalizzati e hanno studiato per dare un contributo al nostro Paese, evitando che siano invece soggetti che che emigrano. Ricordo infatti che siamo interessati da flussi migratori, ma anche da flussi di emigrazione. Vengo da una Regione che ha ancora flussi di emigrazione significativi, pari e anche superiori a quelli dell'immigrazione. soprattutto le nuove generazioni, coloro per i quali abbiamo investito risorse importanti per lo studio e la professionalizzazione; giovani capaci che vanno a giocare le proprie carte da altre parti e che invece noi vorremmo rimanessero nelle nostre comunità, anche in quelle piccole, in maniera tale da sostenere lo sviluppo della nostra terra. Sono questi i temi che dobbiamo affrontare.

il provvedimento di cui oggi discutiamo rappresenta l'ennesimo tentativo del Parlamento di approvare una normativa compiuta per valorizzare i piccoli Comuni. Il testo del disegno di legge infatti, già approvato dalla Camera, ricalca in larga parte le disposizioni del provvedimento che fu approvato nel maggio del 2011 dall'Assemblea di Montecitorio, che purtroppo si arenò subito dopo, proprio in Senato. Prima di ciò furono posti in essere altri tentativi similari sia nel corso della XIV, che della XV legislatura. Quanto detto risulta abbastanza singolare se pensiamo che degli 8.000 Comuni italiani, circa 5.000 di essi hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che insieme rappresentano il 54 per cento del territorio nazionale e nei quali vive il 16,56 per cento della popolazione. Non c'è da stupirsi quindi se le criticità legate alle dinamiche dei piccoli centri nel corso degli anni siano diventate di difficile risoluzione e ampiamente diversificate. L'approvazione del disegno di legge in discussione non è ovviamente in grado di sanare tutte le debolezze e i disagi che affliggono i piccoli Comuni, tuttavia mi auguro possa costituire un'inversione di tendenza da parte del legislatore; un punto di partenza utile per fare chiarezza all'interno di una moltitudine di leggi settoriali che, a vario titolo, interessano le piccole realtà locali. Parimenti, senza un'efficace armonizzazione di tutta la legislazione ad oggi in vigore sulla materia, continueremo ad assistere ad una fallimentare dispersione di risorse economiche e ad una difficile individuazione delle priorità su scala nazionale. Non a caso, i limiti del disegno di legge in esame, sono principalmente due: anzitutto, la previsione dello stanziamento annuo (10 milioni di euro per il primo e 15 milioni dal 2018 al 2023) per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni appare oltremodo irrisoria rispetto alla molteplicità degli interventi che il provvedimento si prefigge di raggiungere. Inoltre, forti perplessità sorgono in merito alle modalità previste per la ripartizione dei progetti da finanziare, soprattutto perché la scelta di accentrare i poteri decisionali a livello governativo rischia di rendere marginale il ruolo delle Regioni che, con il depotenziamento delle Province, sono le amministrazioni che hanno un dialogo più diretto con i piccoli Comuni. Tale condizione apre le porte al problema delle competenze concorrenti tra Stato, Regioni e amministrazioni locali, che verosimilmente potrà rallentare l'esecuzione degli interventi e, quindi, vanificare concretamente lo scopo del provvedimento. Volgendo l'attenzione alle realtà dei piccoli Comuni, appare evidente che il problema principale da risolvere sia quello legato allo spopolamento, dal momento che, senza opportuni interventi, entro i prossimi dieci anni andremo inesorabilmente incontro al rischio di vedere salire al 60 per cento la quota di territorio nazionale abbandonato.

la mancanza di una popolazione numericamente adeguata costringe molte realtà locali a fare a meno di servizi, anche essenziali, per il cittadino. In questo modo, chi se ne è andato non farà più ritorno e coloro che vorrebbero lasciare la vita caotica delle città prediligendo una vita a dimensione umana nei piccoli Comuni sono demotivati proprio a causa della scarsa offerta dei servizi di base. La condizione di marginalità di questi luoghi può essere superata mediante politiche integrate in grado di valorizzare il polo civico di questi territori e per la conservazione delle identità culturali. L'obiettivo che dovremmo prefiggerci di raggiungere come legislatori è quello di creare le condizioni per una politica di crescita economica e sociale dei piccoli centri, in grado di sviluppare i vantaggi della vita civile in tutte le sue forme. Per queste ragioni non va trascurata l'esigenza di avere riferimenti di socializzazione locale volti a migliorare la qualità della vita delle persone residenti; diversamente ci esponiamo al rischio di far diventare i piccoli Comuni delle periferie, luoghi senza identità e senza riconoscibilità. In quest'ottica, i paesi fantasma non sono solo quelli a bassa densità demografica, ma anche quelli che hanno perso la loro specifica cultura e le loro tradizioni, anche dal punto di vista produttivo. Ogni paese o piccolo borgo italiano ha la sua storia da raccontare, anche dal punto di vista produttivo, tanto che il 73 per cento dei borghi più belli d'Italia cento dei piccoli vantano almeno un prodotto con marchio di denominazione di origine protetta (DOP). Sono questi borghi, questi centri storici a rappresentare l'immenso patrimonio nazionale che rende il Belpaese una delle mete turistiche più ambite al mondo. Per questo l'inversione di tendenza cui prima accennavo rappresenta un passo indispensabile per andare nella giusta direzione. Il fatto che il legislatore solo nel periodo compreso tra il 2011 al 2015 abbia operato tagli finanziari ai Comuni per nove miliardi di euro e previsto l'assoggettamento degli stessi alle regole del Patto di stabilità dimostra che un contenimento della spesa pubblica di tipo orizzontale e senza un bilanciamento degli interessi genera enormi disuguaglianze. Interventi che, specialmente nelle piccole realtà, hanno creato forti disagi per le amministrazioni locali. Da questo punto di vista, è necessario mettere in condizione i sindaci e le amministrazioni locali di tornare ad investire sul territorio e non preoccuparsi soltanto di far quadrare i conti. È innegabile che il Governo in questi anni, rispetto alle reali esigenze, abbia concesso molto poco ai piccoli Comuni. Anche questo disegno di legge, senza dubbio animato dalle migliori intenzioni, manca delle risorse economiche per dare seguito alle disposizioni in esso contenute. Il rafforzamento dei piccoli Comuni necessita di interventi multidisciplinari, giacché i caratteri identitari locali possono dirsi preservati soltanto raggiungendo un giusto equilibrio tra le funzioni residenziali, commerciali, del terzo settore, nonché della funzionalità degli spazi pubblici per stimolare la coesione sociale. Il Parlamento deve licenziare definitivamente ancora importanti provvedimenti come il disegno di legge sul contenimento del consumo del suolo, che si pone l'obiettivo di azzerare il consumo di suolo entro il 2050

Pertanto, è necessario prevedere un raccordo normativo, cominciando dalla ricognizione dei provvedimenti già in essere e da quelli che stanno per essere approvati. A maggior ragione quando è difficile reperire risorse finanziarie, queste devono essere utilizzate con intelligenza sulla base di priorità predefinite. L'obiettivo deve essere assicurare la multifunzionalità nei piccoli Comuni, quindi da una residenzialità permanente non rinunciabile, alla promozione di attività produttive, agricole, commerciali e artigianali che siano tra loro interdipendenti. In questo contesto, assume molta rilevanza lo sviluppo tecnologico che, specialmente nelle aree interne e montane fatica a decollare. La realtà, infatti, ci ricorda che ad oggi il 26 per cento dei piccoli Comuni non sono ancora serviti dalla banda larga. Per concludere, c'è ancora molto lavoro da fare per poter ritenere che qualcosa stia realmente cambiando in meglio. Sulla tutela del territorio stiamo ancora muovendo i primi passi. Considerando, però, che da qualche parte si deve pur cominciare, mi piace pensare che l'approvazione di questo provvedimento possa tenere alta l'attenzione su queste importanti questioni per la conservazione dell'incalcolabile patrimonio nazionale che abbiamo ereditato nel corso dei secoli.

a mio avviso assai rilevante, il cui obiettivo è quello di stabilire misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni. Il testo, come è già stato detto, nasce alla Camera dei deputati come Atto Camera 65 del presidente Realacci ed è stato approvato in tale ramo del Parlamento all'unanimità,

Non mi spiego, quindi, i toni dei colleghi della Lega Nord oggi in quest'Aula rispetto al loro voto alla Camera di un anno fa. Anzi, una spiegazione c'è: hanno cambiato idea immagino - all'avvicinarsi dell'appuntamento con le urne. Ma torniamo al provvedimento, perché ognuno risponde dei propri voti ai propri elettori e dovrà spiegare anche queste incongruenze. L'importanza del disegno di legge risiede in particolare nel fatto che questa è forse una delle rare occasioni in cui, a livello istituzionale, viene presa in considerazione una realtà una specifica caratteristica su cui, da sempre, il nostro Paese si basa: i piccoli Comuni, spesso situati in zone interne o in aree montane, in cui milioni e milioni di italiani vivono ed è paradossale che questi cittadini siano spesso assenti nell'agenda politica e istituzionale nazionale. pertanto questo provvedimento un importante passo per invertire tale tendenza. Questa realtà di un gran numero di piccoli Comuni è tipica della Regione dove risiedo, la Lombardia, che conta oltre 1.500 Comuni.

I cittadini che vi risiedono si sentono isolati e, in un certo qual modo, dimenticati. Questa legge segna, mi auguro, una decisa inversione di tendenza. Il testo, dunque, fissa misure per i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi, ciascuno, fino a 5000 abitanti.

inadeguatezza dei servizi sociali essenziali e difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani. In questo provvedimento è possibile individuare tre macro obiettivi: favorire favorire e promuovere lo sviluppo economico-sociale sostenibile, ambientale e culturale dei piccoli Comuni; promuovere l'equilibrio demografico; garantire la tutela e la valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e In tal senso è rilevante l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e incentivare l'afflusso turistico. In tale contesto assumono particolare rilevanza non solo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ma anche quelle di cui all'articolo 8, miranti a incentivare lo sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di *e-goverment*. Più specificatamente il comma 1 dell'articolo stabilisce che le aree dei piccoli Comuni, per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultra larga del 2015, per le aree cosiddette a fallimento di mercato. Non intendo però ripercorrere qui tutti i contenuti del testo, perché è stato già ben fatto dai relatori. Mi limiterò a quelli che mi hanno maggiormente colpito. Grazie alle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Inoltre, nei bandi di gara indetti dai piccoli Comuni, per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva, andrà a costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di tali prodotti, inclusi quelli biologici. Inoltre, i piccoli Comuni potranno destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi ai prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile, con la possibilità per gli esercizi della grande distribuzione commerciale di destinare una congrua percentuale degli acquisti a questi prodotti. La finalità della disposizione è anche quella di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, un obiettivo che andrebbe promosso e implementato a livello non solo locale, ma dovrebbe essere preso come principio guida della politica agroalimentare nazionale. Concludo soffermandomi sull'articolo 15, commi 1 e 2, che prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, il quale deve riferirsi al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. Sono assolutamente favorevole a questa iniziativa, ma avrei auspicato un impegno specifico per il trasporto degli studenti disabili. È innegabile che nei piccoli centri urbani sia ancora più difficile trovare risorse per garantire servizi primari come l'istruzione degli studenti con disabilità. del disegno di legge in esame sarebbe potuta essere un'opportunità per stanziare fondi destinati alla rimozione delle barriere architettoniche, al trasporto degli studenti con disabilità e all'assistenza alla comunicazione per i disabili nelle scuole di ogni ordine e grado. Proprio a tal fine avevo presentato degli emendamenti che però purtroppo - non sono stati recepiti. Si è preferito, comprensibilmente, evitare modifiche al testo per giungere in Assemblea alla sua approvazione definitiva. Confido però che nella prossima legge di stabilità si possa rimediare a questa mancanza, incrementando il fondo creato dall'articolo 3 del provvedimento. Concludo davvero augurandomi che il provvedimento in esame non solo venga approvato, ma che sia davvero il primo passo di un percorso di maggiore attenzione alla realtà dei piccoli Comuni.

ho pensato che ci fosse un errore di stampa, un refuso. Quando ho letto la cifra di 10 milioni ho pensato che mancasse qualche zero, perché in tutti gli articoli di cui il disegno di legge si dipinge in modo chiarissimo qual è lo scenario dei bisogni del territorio. L'Italia è fatta di una somma di territori, non è una nazione

euro ad abitante per dieci anni vuol dire un euro all'anno. Facciamo un confronto con le cifre stanziate per il finanziamento per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese:

Questo è denaro fornito dai contribuenti. Ricordo che i contribuenti sono tutti gli italiani: un insegnante che vive in un piccolo Comune è contribuente esattamente tanto quanto un insegnante che vive in una grande città.

chiederanno conto. Infatti, questa è una Repubblica in cui - giustamente - per ogni cittadino c'è un voto. Questa politica, che è non solo di questo Governo ma degli ultimi vent'anni, ha manifestato la sua totale incapacità di ricongiungere due realtà: la realtà che piace accarezzare, quella che adesso vorrei rappresentare con l'esempio dei grandi poli museali

importante di necessità e idee per la valorizzazione che vengono finanziate con un euro per abitante al giorno. È uno schiaffo!

all'articolo 3, dove si inserisce questo fondo, è scritto che, per quanto possibile, verrà assicurata un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. «Per quanto possibile»? Ma come? E soprattutto verrà data priorità al finanziamento degli interventi proposti da Comuni istituiti a seguito di fusioni o appartenenti a un'unione di Comuni. Questa, quindi, è la vera finalità del provvedimento: spingere verso

di una burocrazia ragionieristica di mezze maniche che stanno sedute davanti ai loro conti e, senza guardare alla realtà del nostro Paese, si preoccupano di fare un ragionamento di tipo contabile. La fusione e l'unione dei Comuni, già resa difficile da una storia e una cultura che vedono il loro pregio e il loro valore nella differenza,

alla realtà del nostro territorio e di essersi invece arroccati sulla ricerca di un consenso su grandi agglomerati, che ha fatto perdere di vista la nostra vera ricchezza; ora, però, però, si pretende da parte dei piccoli Comuni uno sforzo che va non solo contro la loro cultura, ma anche contro le loro oggettive capacità di condividere servizi. Questo è l'insulto più grosso.

anzi, viene chiesto di corrispondere agli stessi obblighi che vincolano i grandi Comuni, senza avere le risorse né il personale.

si pretende di assegnare questo denaro sulla base di bandi. Non sono affatto d'accordo con l'opinione espressa da diversi colleghi che salutano il concetto di bando come un omaggio alla meritocrazia, perché stiamo parlando di bisogni. Il bando è comprensibile quando si hanno davanti soggetti, per esempio le aziende, che giustamente devono essere messe alla prova sulla loro capacità di

umane necessarie per costruire quei bandi. Si chiede ai Comuni di investire magari in società private che allestiscano i bandi Se io sono lo Stato e raccolgo denaro dai contribuenti per distribuirlo sul territorio, non lo faccio sulla base del merito dei singoli cittadini del territorio ma sulla base dei bisogni. Una località che

Per esempio, abbiamo parlato del servizio postale. Sono stati chiusi alcuni uffici postali nelle aree periferiche perché bisognava realizzare economie di scala. Le economie di scala, però, non possono essere messe in campo se producono un danno e quindi una minore possibilità per determinati cittadini di usufruire di un servizio che deve essere ovviamente uguale, come abbiamo già detto, a quello

il decreto legislativo n. 504 fu introdotto il Fondo nazionale speciale per gli investimenti che finanziava, con i proventi del casinò di Campione d'Italia, gli interventi che dovevano essere fatti

11 milioni di euro del 1996 non sono ovviamente 10 milioni di euro del 2017; quindi mi sembra che siamo arretrati rispetto a ciò che facevamo vent'anni fa. fa. Questa è un'evidenza del fatto che le somme messe a disposizione sono veramente ridotte. D'altra parte, dobbiamo ricordarci sempre dell'articolo 3, dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che mi permetterò di leggere: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Noi dovremmo allora andare in questa direzione. Come potremmo fare? Ci sono questioni che riguardano la banda ultra larga, un tema a me particolarmente caro. caro. Dobbiamo far sì che una persona possa utilmente lavorare, soprattutto in un'area lontana dai centri urbani; con le tecnologie disponibili tramite la rete, questo si può fare. Ci sono quindi questi aspetti, che sono sicuramente molto interessanti, anche perché le aree dei piccoli Comuni che ricadono nei *cluster* D, dove cioè nessuna azienda ha intenzione di intervenire e quindi interviene lo Stato,

è una cosa utile, sempre che non si tolgano gli sportelli di prossimità. L'efficienza e l'economicità della pubblica amministrazione non devono essere realizzate a scapito della possibilità, per l'utente che vive in un piccolo Comune, di avere uno sportello di prossimità. Questo va bene.

Pertanto, quando parliamo delle persone che vivono in questi Comuni,

Non c'è bisogno che vi ricordi la canzone che diceva: «Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città». Era Giorgio Gaber, tantissimi anni fa,

Quando parliamo del piano generale dei trasporti, che deve connettere meglio i piccoli Comuni, va bene, ma bisogna vedere come verrà coniugato. Quando parliamo, ad esempio, del fatto

Anche qui potrei citare Gaber quando diceva che l'idea è come un gabbiano ipotetico, ma poi il sogno si è rattrappito. è rattrappito. Bisognerebbe avere il coraggio di volare un po' più in alto, di riuscire a far sì che le cose che vogliamo mettere in campo siano potentemente forti. Solo con un'azione spinta e risoluta potremo contrastare la dinamica che ci porta tutti ad essere iperproduttivisti per rimettere al centro l'uomo e la nostra capacità di essere uomini e non macchine. Questo è un primo passo, però si può e si dovrebbe fare di più. Mi auguro che nella prossima legislatura riusciremo a fare quel passo definitivo che non siamo stati in grado di fare in questa.

significa meno di 2.200 euro all'anno per ciascun Comune. Se calcoliamo che ogni immigrato che arriva con i barconi costa allo Stato, una volta arrivato e salvo spese straordinarie, 2.200 euro al mese, vuol dire che un immigrato vale quanto 12 piccoli Comuni ai sensi di questa legge. come dicevo, sono sempre meglio 15 milioni all'anno che niente, anche se siamo molto vicini al nulla. Faccio un altro paragone. Il Fondo di solidarietà fra i Comuni, bizzarra istituzione, fa sì che i Comuni virtuosi debbano tirare fuori dei soldi per i Comuni non virtuosi. È un sistema assai discutibile, ma per lo meno dovrebbe essere tra Comuni:

ai piccoli Comuni. Non so se rendo l'idea di quali dimensioni stiamo parlando. La questione dei piccoli Comuni è stata fatta oggetto di gran parlare: «bisogna ridurre gli sprechi!». Ricordo al Movimento 5 Stelle che nel suo programma del 2013, quello con il quale sono stati eletti i colleghi presenti al Senato e naturalmente anche nell'altro ramo del Parlamento, comprendeva l'accorpamento dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, perché, a quanto pare, i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono uno spreco.

i Comuni tutti, dal più grande al più piccolo, devono fornire una serie di servizi ai cittadini. In generale, se parlassimo di aziende, effettivamente, per l'economia di scala, dovremmo immaginare che i Comuni grandi forniscano servizi a costo inferiore, per una duplice ragione: perché sono più grandi (è la famosa economia di scala) e poi perché hanno, nella grande maggioranza, un territorio più semplice da governare. Per fornire un servizio a centomila milanesi, a centomila romani, a centomila torinesi, vi è un territorio, intanto pianeggiante (forse a Roma un po' di meno), dove

di spettanza dei Comuni, spendono circa 1.578 euro *pro capite*, mentre la media generale è di 938 euro. Ma guarda un po': sono i Comuni più grandi quelli che spendono di più. Al secondo posto per spesa elevata e, dunque, per cattiva gestione o, comunque, per maggiori costi nel fornire questi servizi vi sono i Comuni fra i 60.000 e i 250.000 abitanti, cioè la seconda fascia più alta per popolazione dove, comunque, siamo ancora sopra la media. I Comuni sotto i 60.000 abitanti mediamente hanno costi inferiori. I Comuni sotto i 5.000 abitanti, che hanno tutte le difficoltà che ho descritto prima (pochi abitanti sparpagliati su un territorio esteso, per cui nessuna economia di scala e notevoli disagi territoriali), sono ben sotto la media, circa il 10 per cento sotto la media di spesa. Ma allora come mai bisogna massacrare i piccoli Comuni? Da Da qualche anno, ai grandi mezzi di informazione e ai partiti politici che li seguono piace accorpare, uniformare e omologare. Questo alla faccia dell'articolo 5 della Costituzione che vanta

è mai cambiato, alcune leggi che hanno fatto esattamente il contrario, senza neppure realizzare risparmi di spesa. La soppressione di tanti tribunali e uffici giudiziari

risparmio è stato pari allo zero assoluto. Si era promesso un risparmio vicino allo zero, di 80 milioni in tre anni, ma il risparmio è stato zero. Se ne è accorto anche il Partito Democratico che aveva nel suo programma del 2013 il ripristino di alcuni tribunali, elencati per nome (cito quello di Pinerolo perché si Regione, ma ve ne erano altri). Tutti gli emendamenti da me presentati, che riproducevano, parola per parola, il programma del Partito Democratico, hanno ricevuto parere contrario e sono stati respinti dalla maggioranza di quest'Assemblea. Poi, però, si fa la leggina dei piccoli Comuni. La legge Delrio ha massacrato le comunità locali: avendo reso le Province un ente disarticolato, senza risorse, lontano dai cittadini, ha scoraggiato perfino gli unici a cui è rimasto il diritto di votare alle elezioni provinciali,

prima o poi lo fanno; se non lo vogliono fare, vi sarà anche una qualche ragione, visto che riescono ad avere costi inferiori a quelli dei grandi Comuni che dovrebbero prendere ad esempio. dopo aver ottenuto un paio di proroghe, la norma è entrata in vigore. Il risultato è che la stessa burocrazia che grava sui grandi Comuni grava sui piccoli Comuni, con l'aggiunta di un problema: una volta che il Comune ha i soldi e ha ricevuto tutte le autorizzazioni

la riduzione dei centri di spesa vale sempre lo stesso criterio. Credo sia importante ridurre la spesa, e non i centri di spesa, specialmente in un Paese in cui l'articolo 5 della Costituzione parla del più ampio decentramento amministrativo. Concludo dicendo cosa servirebbe ai piccoli Comuni e che non costa niente, anzi sarebbe un risparmio per lo Stato: meno burocrazia. Se parlate con i sindaci, vi diranno negli ultimi cinque anni il lavoro per fare le stesse cose che si facevano in passato è aumentato del 30-40 per cento; 30-40 per cento di lavoro in più per fare le stesse cose di cinque anni fa. Il tutto avviene - come dicono le leggi - senza maggiori spese. Certo, ma ciò vuol dire che puoi offrire meno servizi ai cittadini:

gli incarichi per i dipendenti e, quando un Comune ha un solo dipendente, deve fare una lunga relazione in cui deve spiegare come mai non ha fatto la rotazione degli incarichi), i piani della trasparenza, i piani delle *performance* e altre cose.

i ceti mercantili, le arti e i mestieri, i piccoli e medi borghesi si organizzano e prendono in mano la gestione della municipalità,

l'istituzione del Comune, che poi viene esportata in tutto il mondo. L'istituzione della municipalità e del Comune è croce e delizia dell'Italia, perché spesso siamo affetti da municipalismo; spesso le diatribe tra Comuni e municipalità fanno premio sulle sinergie che sono state anzi tempo evocate, ma sono una delizia perché rappresentano la radice del nostro essere, la vera radice dell'Italia. È vero che la Costituzione dice che l'Italia si divide in Comuni, Province e Regioni, ma è vero pure che il 99 per cento degli italiani sentono la loro radice, il loro essere nell'appartenere a un determinato Comune o a un altro.

omettono di dire che, oltre ai 100 milioni di euro stanziati nel testo, il provvedimento consente di rientrare all'accesso di 2,2 miliardi di euro stanziati dal CIPE nel 2015 per i Comuni delle cosiddette zone zone bianche. A me non piace utilizzare la definizione europea di zone economicamente a fallimento, ma comunque si tratta delle zone in cui gli operatori privati - ci rientrano il 99 per cento dei piccoli Comuni - non hanno interesse a investire. Il CIPE nel 2015 - non nel 2008 o nel 2009, mi dispiace, senatore Malan - ha stanziato 2,2 miliardi di euro e i bandi

L'articolo 9 incentiva l'apertura e la non chiusura degli uffici postali e ricordo anche - lo dirò martedì prossimo in un'audizione all'amministratore delegato delle Poste - che la convenzione e il decreto ministeriale del 2008 vieta alle Poste di chiudere uffici postali in piccoli Comuni e definisce come servizio postale universale la copertura di almeno il 96 per cento dei Comuni italiani.

ho citato infatti prodotti e valori che ci sono, che producono economia - e che quindi va tutelata nelle forme e nei luoghi più opportuni.

della riparametrazione delle indennità degli amministratori dei piccoli Comuni. Fare oggi l'amministratore nei piccoli Comuni è sostanzialmente un'opera di volontariato. Negli anni abbiamo ridotto talmente tanto le loro indennità e la loro possibilità di prendere permessi, che sostanzialmente sono arrivate ad alcune decine di euro al mese.

sono persone che hanno dovuto prendere dei permessi dal lavoro e perdere indennità di lavoro, perché non hanno possibilità di poter esercitare in maniera dignitosa la riparametrazione a livelli di sussistenza economica delle indennità degli amministratori dei piccoli Comuni non è un tema molto popolare in un momento in cui culturalmente, di alcuni movimenti politici, ma anche di alcuni giornali, viene assaltata l'idea che componenti dell'amministrazione e della politica debbano avere un'indennità. Anzi, si dovrà arrivare al punto in cui dovranno esserci delle sanzioni economiche

ma, soprattutto, è una bella giornata per l'Italia.